L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunico che, d'intesa con la Camera dei deputati, le Commissioni parlamentari bicamerali - della cui composizione è stato dato annuncio nella seduta del 19 luglio scorso sono convocate, per la loro costituzione, domani, giovedì 25 luglio, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario, secondo i seguenti orari: - ore 8,45: Commissione enti gestori; Commissione infanzia e adolescenza; Comitato Schengen; Commissione anagrafe tributaria. - ore 14 : Commissione questioni regionali; Commissione semplificazione. Comunico inoltre che, sempre nella giornata di domani, sono convocate, per la loro costituzione, le delegazioni presso le Assemblee parlamentari NATO, Consiglio d'Europa, INCE e OSCE, secondo i seguenti orari: ore 8: Delegazione Assemblea parlamentare NATO, presso il Senato della Repubblica, Aula piano terra, Palazzo Cenci; - ore 14: Delegazione Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, presso la sede di Palazzo Valdina, sala Soprachiesa; - ore 14,45: Delegazione Assemblea parlamentare INCE, presso la sede di Palazzo Valdina, sala Soprachiesa; - ore 15,30: Delegazione Assemblea parlamentare OSCE, presso la sede di Palazzo Valdina, sala Soprachiesa.

Presidente, anch'io desidero segnalare che ero regolarmente al mio posto, ma non ho recuperato in tempo la tessera che mi hanno fornito cortesemente, ma purtroppo in ritardo.

il presidente Gasparri ha ritenuto di affermare: «Mi auguro che tale rinvio consenta di affrontare questo delicato provvedimento in condizioni migliori di quanto non sia stato fatto finora». Orbene, poiché ricordo con quanta pazienza il presidente Gasparri nella precedente legislatura ebbe a seguire i lavori relativi al disegno di legge sulla diffamazione, ritengo che questa non sia una simpatica tirata di orecchie, ma un monito a considerare conclusa la fase di rodaggio che caratterizza questa maggioranza di larghe intese, così dicendo in chiaro la ragione per la quale avevo chiesto l'aggiornamento della seduta e il rinvio al giorno successivo.

il 3 luglio la Commissione affari costituzionali ha rilasciato il prescritto parere sui presupposti di costituzionalità. I lavori sono iniziati in Commissione il 9 luglio, concludendosi la discussione generale, articolata e complessa, il successivo 16 luglio.

Prima di darle una risposta, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione sui nuovi emendamenti. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.520, 2.800, 2.170, 2.180, 3.1000,

procedurali che incidono negativamente sulla reale concretizzazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione.

il parere sull'ordine del giorno G2.100 è contrario.

carceri che strutturalmente non sono idonee. L'emendamento dispone che se l'istituto penitenziario presso il quale il condannato deve scontare la pena detentiva è fatiscente, o comunque non conforme alle norme di

Vi sottopongo queste riflessioni perché sono naturali: non possiamo dire di no a tali evidenze.

ovviamente non illustra, perché si tratta di questione già trattata.

si propone che non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. questo caso, la considerazione relativa alla necessità di garantire - da una parte - i problemi attinenti alla sicurezza sociale e - dall'altra - salvaguardati questi problemi, di consentire al tossicodipendente di proseguire il programma terapeutico di recupero, soprattutto nel caso in cui l'interruzione possa pregiudicarne lo stato di salute. Naturalmente - la parte finale dell'emendamento va proprio in questo senso - se esistono strutture idonee presso le strutture carcerarie,

due emendamenti fondamentali: prima di tutto l'emendamento 4.9, relativo alla questione del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie.

la possibilità di reinvestire i proventi delle dismissioni degli istituti e degli immobili carcerari in nuove strutture carcerarie. Questo, allo stato e così come è scritto l'emendamento (impegnandomi insieme ai colleghi eventualmente a riscriverlo in un prossimo provvedimento) viola esplicitamente

riduce gli obiettivi del debito e deve coprirli. Noi invece riteniamo possibile, attraverso una adeguata interlocuzione, così come è stato già fatto, superare il problema, e ci impegniamo a farlo. Pertanto, per il momento rimane la nostra contrarietà in base all'articolo 81.

sapendo che è difficile che l'amministrazione pubblica riesca a metterla immediatamente, e questo per coprire una spesa strutturale permanente e crescente, di natura corrente. Per questo motivo rimane la nostra contrarietà su questo punto. Voglio sollecitare tutti i colleghi a capire che quando si parla di spesa per il personale dobbiamo trovare forme di copertura che abbiano un adeguato livello di capienza, ma anche un elevato livello di liquidità, perché è ovvio che la spesa corrente per il personale è quella in cui cassa e competenza si avvicinano

a prescindere dalla nostra azione, che magari può anche essere intesa come ostruzionistica, chiedo ai colleghi se non sia il caso che la Commissione si riunisca, dopo aver fatto in quella sede le votazioni, come detto dal presidente Palma, in tutta fretta per arrivare in Aula, e faccia una

dicano. Non è possibile che il relatore, a prescindere dalla Commissione, si prenda la responsabilità continuativa di modificare in maniera assolutamente incisiva gli emendamenti della Commissione stessa. *(Applausi dai

commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o contro la persona"».

perplessità in quanto è in piena coerenza con l'impostazione e con l'idea che emerge dal decreto-legge. Intanto di chi parliamo? Parliamo di persona tossicodipendente o alcoldipendente

deve aver commesso un reato connesso alla sua condizione specifica di tossicodipendente.

Quindi c'è una clausola di garanzia, rispetto al controbilanciamento sulla necessità di mantenere in piedi il percorso terapeutico, verso la condizione di sicurezza e di garanzia per i cittadini che non ci sia un uso arbitrario di questa condizione o un aggiramento della stessa per non subire i rigori della custodia. custodia. Di fronte a un emendamento così congegnato, che è in grado di bilanciare l'intervento terapeutico con il rigore e e con una condizione che evita qualunque aggiramento, penso che questa sia la filosofia complessiva del decreto, che apre alla custodia cautelare, che apre alla detenzione detenzione domiciliare, senza che questo pregiudichi la domanda di sicurezza che è presente nel nostro Paese. Questo è un caso

dice che un soggetto tossicomane o alcoldipendente - inserendo una nuova tipologia rispetto ai trattamenti di favore già previsti dalla legge con riferimento ai tossicodipendenti o agli assuntori di sostanze stupefacenti, sostanzialmente gli alcoldipendenti

disponibili strutture carcerarie idonee alla prosecuzione del programma in corso, vale a dire sempre.

un soggetto tossicodipendente o alcoldipendente che, ad esempio, travolge e uccide tre persone ipotesi sufficientemente frequente, tant'è vero...

il legislatore di recente ha modificato il reato di omicidio colposo prevedendo un'aggravante ad effetto speciale quando l'omicidio colposo si correla all'uso e all'abuso delle sostanze stupefacenti o alcoliche - a meno che il giudice non intraveda

Quali sono le esigenze cautelari? Pericolo di fuga? Dubito vi possa essere. Esigenze di inquinamento delle prove? Il fatto c'è, la macchina ha travolto tre persone, non vi è un problema di inquinamento probatorio. Inoltre la possibilità di reiterazione dei reati dei reati deve essere necessariamente esclusa in ragione del programma di recupero a cui il soggetto è sottoposto. Sostanzialmente, attraverso questa norma creiamo una categoria di soggetti per i quali la custodia cautelare non potrà essere applicata. Signora Presidente, intervengo per richiamare i colleghi alla delicatezza estrema della materia. Personalmente sono sempre stato favorevole al fatto che i tossicodipendenti vengano recuperati nelle comunità di recupero, dai SERT, SERT, senza essere incarcerati. Ma faccio presente che già esiste una normativa che prevede, per le condanne fino a sei anni di carcere (anche con sentenza passata in giudicato), la possibilità di espiare la pena presso comunità di recupero o presso strutture pubbliche.

proprio per poter raccogliere dei suggerimenti pervenuti all'interno della Commissione da senatori di vari Gruppi politici, tra cui ricordo il senatore Caliendo.

l'articolo nella sua interezza. Quando, infatti, si parla della impossibilità di disporre la misura della custodia cautelare in carcere si fa riferimento alle persone che abbiamo indicato,

quando facciamo salve le esigenze cautelari, facciamo espressamente riferimento a tutte e tre le esigenze, tra cui quella ricordata dal presidente Palma alla possibilità di reiterazione del reato. Sussistendo la possibilità di reiterazione del reato è chiaro che non si procede all'indicazione che noi diamo. Siccome si tratta di situazioni molto delicate e sensibili che riguardano delle persone, che hanno certamente dei problemi di tossicodipendenza o di alcoldipendenza e che, peraltro, bisogna tutelare da loro stesse, come bisogna tutelare anche la comunità da eventuali loro comportamenti, credo che gli scrupoli che abbiamo avuto nell'indicare tutti questi passaggi

dopo le parole "«e 3-*bis*»" delle seguenti: "e le parole «sulla base delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse»". Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi».

4.6 è riferito alla veste di immobiliarista di questo commissario. Non mi sembra il caso che si vadano a fare operazioni lucrose riguardo apparati edilizi mentre ci sono una serie di edifici già costruiti che potrebbero essere utilizzati. Quindi, prima di pensare a nuove costruzioni, andiamo a recuperare quelle esistenti.

Signora Presidente, alla luce di quello che ha affermato il presidente Azzollini, che ringrazio per il suo intervento, la Commissione ritira l'emendamento 4.9 credo che, di conseguenza, venga a cadere anche l'emendamento 4.9/3 del senatore Caliendo, sia nella prima che nella seconda formulazione.

Con questi emendamenti e ordini del giorno noi vogliamo favorire quello che nel Paese non siamo mai riusciti a fare. Noi abbiamo un'unica garanzia: per costruire un carcere ci vogliono più di vent'anni. Ieri avevo sottolineato il fatto che talvolta la parte politica e la parte amministrativa riescono a fare sintesi nel Paese, ovverosia riescono a trovare un accordo serio e concreto per la costruzione di un carcere. Ho portato ad esempio il caso del Comune di Milano, in cui l'allora sindaco Albertini e l'allora ministro Castelli trovarono una soluzione per la questione di San Vittore, creando veramente un'idea e un progetto di eccellenza. Cos'è successo? Come spesso accade nel nostro Paese, si è alzato una mattina un provveditore, in questo caso alle opere pubbliche

sanitaria attuale. Quindi, poiché abbiamo a cuore la sanità penitenziaria, almeno per la parte della messa a norma dei locali che saranno messi a disposizione delle ASL a seguito del passaggio previsto dal decreto del

(se possono funzionare le piccole carceri), anche se era pleonastica per alcuni di noi che conoscono la realtà carceraria. Le piccole strutture carcerarie non sono idonee a garantire procedimenti e trattamenti corretti e, dall'altro lato, comportano un impegno di Polizia penitenziaria che è scombinato rispetto all'organizzazione generale. va per legge a stabilire una certa procedura, quando invece essa va verificata in concreto. La risposta del Ministro è stata che, con meno di 250 detenuti, qualsiasi struttura carceraria non è in condizione

un incontro collettivo con gli psicologi a cui ho partecipato anch'io due volte per due ore. È quella la funzione che noi dobbiamo recuperare.

dell'organizzazione carceraria la valutazione in ordine a quando è proprio necessario mantenere una struttura che non risponda ai criteri di efficienza di cui ha parlato il Ministro.

che sulla individuazione delle piccole strutture carcerarie, sostanzialmente quindi sui criteri di economicità, vi è stato un approfondimento e il ministro Cancellieri specificato che secondo i parametri del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria una struttura carceraria viene considerata economica

per differenziare dobbiamo evitare che la ristrutturazione di cui ha bisogno il circuito carcerario faccia l'errore di concentrare tutto sui grandi poli.

per trovare una soluzione, perché accogliere come raccomandazione un ordine del giorno che dice la stessa cosa di un emendamento

rimanere in questo ambito, senza un impegno ulteriore rispetto a ciò che il Parlamento ha fatto, rappresenti un punto di equilibrio utile per tutti. Signor Presidente, vorrei chiarire i termini della questione. Noi abbiamo approvato un emendamento, il cui contenuto è sostanzialmente questo: il Commissario riferisce ogni anno sull'attività svolta, e, con riferimento all'anno in corso, riferisce entro il 31 dicembre. Quindi, i parametri delle risposte e delle informative del Commissario sono chiariti per legge.

i parametri con cui il Commissario deve informare il Parlamento. Se l'ordine del giorno in questione è in linea con quell'emendamento

con l'emendamento 5.200 si chiede di inserire una norma di salvaguardia dei finanziamenti attuali per i programmi terapeutici e di recupero concernenti le persone tossico o alcoldipendenti detenute, in quanto nell'annualità 2006, a seguito dell'indulto, i fondi a disposizione furono ridotti di una percentuale proporzionalmente pari ai detenuti che beneficiarono dell'indulto. Successivamente, ed anche abbastanza rapidamente, la popolazione detenuta registrò un nuovo incremento ma i fondi rimasero sostanzialmente invariati.

già stanziati, quindi non ci sono aumenti. Vuol dire che pensiamo di tagliare retroattivamente i fondi già stanziati sulle tossicodipendenze? Sono portata a pensarlo. Mi pare che siamo già messi abbastanza male

l'esigenza dell'Aula e i doveri della 5a Commissione affinché venga risolto il problema della sindacabilità o dell'insindacabilità dei pareri della stessa, che noi rispettiamo, per carità, nel modo più categorico. pare però che il gesto della collega Granaiola sia cortese: non è un atteggiamento ostruzionistico in quanto premette la disponibilità a ritirare l'emendamento; si chiede soltanto di conoscere, di fronte ad un emendamento,

in una prossima seduta può risolvere questo problema, credo che avrà anche risolto in generale una situazione di amarezza

uno spirito preciso. Se così non fosse, però, mi stupirei di tutti voi, colleghi, perché parliamo di diritti ma nel momento in cui dobbiamo confermare

termine - quando dobbiamo sottostare alle indicazioni della Commissione bilancio (che, per carità, fa il suo mestiere), ma ci sono degli elementi di principio che secondo me vanno mantenuti, e questo è un emendamento che va mantenuto.

e quindi non sono a riserva, ma rientrano nella contabilità pubblica. A questo punto dovremmo rivedere il bilancio dello Stato e non siamo in condizioni di farlo e avremmo evidentemente, in taluni casi, un aumento di spesa, in altri un'invarianza di spesa.

In realtà ci atteniamo al fatto che, nel momento in cui dei fondi avanzano o sopravvengono, non esistono parti di competenza del bilancio che riservano quei fondi al Ministero della sanità piuttosto che alla tal Regione o al Ministero della difesa:

rispetto all'invarianza di bilancio, fermo restando che se esso non determinasse nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ciò francamente mi tranquillizzerebbe dal punto di vista del bilancio.

pensa di utilizzare le risorse destinate al recupero dei tossicodipendenti per finanziare questo decreto.

senatore Buccarella,

la lettera dell'emendamento stesso non sembra far temere aumenti di spesa. Infatti nell'ignoranza di chi vi parla, leggere che sono fatti salvi i finanziamenti attuali per i programmi terapeutici e di recupero e, a seguire, e, a seguire, il testo dell'articolo 5, in cui è stabilito chiaramente che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non credo possa

di quest'Aula. Mi spiace, naturalmente, dover andare forse contro un nobile motivo, ma se così fosse ogni volta ci incarteremmo

anzi la certezza, che il provvedimento poi venga restituito alle Camere dal Quirinale per palese incostituzionalità, data la violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Quindi, vorrei invitare i colleghi a

Signor Presidente, intanto ringrazio moltissimo il senatore Sangalli che ha dato una motivazione plausibile e

comunque, il punto di soldi che non sono stati spesi. Io chiedo, pertanto, che il Ministro competente venga in Aula a spiegare perché i fondi non vengono utilizzati.

e qui scopriamo, belli belli, che ci sono dei fondi non utilizzati per far fronte ad un tema drammatico! Quindi, chiedo ufficialmente, signor Presidente, di avere qui in Aula quanto prima il Ministro competente per spiegare. Detto questo, non credo sia possibile dividere l'Aula su un tema socialmente sentito da tutti, ma che confligge con una norma rispetto alla quale - ahimè - non si può dire nulla. Quindi, propongo alla senatrice Granaiola, e agli altri sottoscrittori

Presidente, anch'io ringrazio il senatore Sangalli, ma, ahimè, non mi ha convinto, e quindi permane la mia totale contrarietà,

i colleghi, quando sottoscrivono un emendamento altrui, usare la formula «faccio proprio» o «faccio mio» l'emendamento del collega. Molto sommessamente, ritengo allora che questa espressione

Sul punto ne approfitto, in qualità di cofirmatario, chiedendo che l'emendamento vada ai voti. In più sottolineo che quello che sta succedendo in questi minuti è la rappresentazione plastica, visto il riferimento all'articolo 81 della Costituzione e ai vincoli che nel 2012 lo Stato italiano ha assunto, forse in maniera troppo frettolosa,

il non aumento delle spese pubbliche, quando nel caso concreto - nell'ignoranza di chi sta parlando - non mi pare che sia astrattamente ipotizzabile un maggiore impegno di spesa, è la rappresentazione plastica di come la decretazione d'urgenza - ma di questo parleremo dopo - e gli obblighi di asservimento dello Stato italiano alle politiche monetarie europee, con il *fiscal* *compact* e tutto il resto (che ha comportato la modifica estiva e balneare dell'articolo 81 della Costituzione), ci mettono in difficoltà anche quando parliamo di

Costituzione non è un colpo di Stato: è semplicemente una norma che prevede una gestione ordinata del bilancio, in cui le poste attive e le poste passive siano chiare. Non ci possono essere poste attive di presunti avanzi, perché gli avanzi di amministrazione entrano nel generale *stock* di debito che abbiamo; non possiamo separare le diverse parti dello Stato dal bilancio unitario dello Stato. Per tutto questo, la Commissione bilancio

in cui si dice che, conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine giorno, ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento, gli altri firmatari non possono chiedere la votazione dell'emendamento. Prendiamo atto di questo parere e agiamo di conseguenza.

punto, o la Commissione bilancio dice che, in assenza di questi fondi, non vi è la copertura dell'articolo 5, ovvero non riesco a comprendere davvero la ragione, ove le risorse finanziarie nel bilancio generale vi dovessero essere, per la quale noi qui non possiamo affermare che nel reperimento delle risorse finanziarie vi è un ostacolo con riferimento esattamente a quei fondi che sono attualmente utilizzati per il recupero dei tossicodipendenti. Se si dovesse accedere all'interpretazione che io sommessamente propongo (le risorse finanziare sono quelle del bilancio, trovatele dove vi pare ma non potete utilizzare questi fondi), il problema è un altro, in tutta la restante parte del bilancio vi sono o no le risorse finanziarie. Si tratta semplicemente di un ordine prioritario nell'individuazione delle risorse finanziarie e di un'esclusione

desidero ringraziare il relatore, senatore D'Ascola, tutti i componenti della Commissione giustizia, i funzionari, dottor Martinelli e dottoressa Annecchiarico, la dottoressa Andreuccioli e tutto il personale della Commissione per per l'eccezionale lavoro che hanno svolto nei ristretti tempi consentiti alla Commissione per poter arrivare in Aula e consentire, a seconda della votazione finale, la definizione di questo provvedimento.

Ne vengono elogiati i meriti e gli atti eroici, eppure appartiene ad un settore che negli ultimi cinque anni ha subito un taglio ai finanziamenti di 3 miliardi di euro, un taglio alle assunzioni del 50 per cento e a cui sono stati detratti 721 milioni di euro dagli stipendi 2012-2013. depauperata a tal punto che certi uffici funzionano solo grazie al fatto che i lavoratori si comprano la carta per le stampanti. Pensate, noi abbiamo quella filigranata. dove, se si viene promossi dopo anni, si prende meno di quando si era al grado inferiore. Sto parlando di chi, in queste condizioni, deve garantire la sicurezza del Paese, di chi in queste condizioni serve lo Stato: sto parlando della polizia e dei poliziotti. Non voglio parlarvi di quando vengono schierati a fronteggiare la rabbia dei lavoratori o dei disoccupati o di quando i Governi, presenti e passati, li rinchiudono in fortini Il vero problema per questi, come per tanti altri lavoratori, sono i politici e i Governi che hanno fatto tante promesse e non le hanno mai mantenute; sono l'ingerenza nelle nomine di funzionari politicizzati e le ingiustizie. Quei poliziotti che onestamente e con dedizione svolgono il loro lavoro e garantiscono la nostra sicurezza sono stanchi.

i cittadini aspettano ore per fare una denuncia. Infine, senza lavoro e senza la pace sociale, le piazze saranno sempre più piene. Lo scenario è questo e di questo passo peggiorerà.

Signor Presidente, egregi colleghi, chiedo l'attenzione dell'Aula per manifestare il mio ringraziamento alle forze dell'ordine, per il lavoro importante che svolgono quotidianamente tra mille avversità,

ha sentito quattro colpi di fuoco provenienti dall'esterno e, contemporaneamente, delle grida di persone impaurite da quello che stava accadendo. accadendo. Immediatamente Rita Scopelliti, in tutto questo disarmata, si è avviata verso l'esterno della chiesa mettendo in sicurezza alcune persone presenti sulla via Arangea, luogo dei fatti, e facendole riparare dietro automobili in sosta, contattando contestualmente la sala operativa del 113. La poliziotta, inoltre, è accorsa senza esitare verso una donna ferita e chinata per terra, purtroppo poi deceduta, ed altre due persone, tra cui un ragazzo, per proteggerle dall'aggressore. Infine, Rita Scopelliti intercettava un uomo anziano, di circa settant'anni, il quale era stato individuato come l'autore degli spari e lo consegnava agli agenti nel frattempo intervenuti. Signor Presidente, colleghi senatori, permettetemi di esprimere in quest'Aula il mio sentito ringraziamento a Rita Scopelliti, donna che opera al servizio dello Stato con umiltà e senso di responsabilità, per l'immediato intervento azionato, che ha scongiurato ulteriori fatti sanguinosi. Consentitemi altresì di rivolgere un apprezzamento per l'azione che le forze dell'ordine della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza e tutti gli apparati di controllo svolgono giornalmente per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Considero tali gesta meritevoli di menzione, perché come cittadino di questo Paese e come senatore della Repubblica sento il dovere personale, nonché istituzionale, di esprimere il mio semplice ed umile compiacimento per quanto accaduto,

Ricordo che alla città di Roma è stata conferita la medaglia d'oro alla Resistenza e che chi vuole festeggiare un criminale di guerra si rende partecipe di una grave responsabilità. Erich Priebke è stato condannato all'ergastolo perché ritenuto tra i responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine: onorare il boia di quella efferata strage significa offendere la memoria delle vittime del nazifascismo, che mai dobbiamo dimenticare.

perso la vita in giovane età. Un carnefice non può essere mai festeggiato e le ragioni della giustizia e della verità storica non possono essere oscurate. A nessuno è consentito di assolvere la barbarie nazifascista e screditare la Resistenza, che fu alla base della nascita della Repubblica e del ritorno alla democrazia. L'omaggio a Erich Priebke, che da alcuni giorni personaggi più o meno noti annunciano di voler fare, è una strumentalizzazione politica inaccettabile, sulla quale le istituzioni, senza alcuna deroga, debbono vigilare per impedire qualsiasi atto di ossequio privato o pubblico verso chi non avrebbe meritato alcuna indulgenza da parte dello Stato italiano. Nell'esprimere solidarietà alle famiglie dei martiri, molte delle quali ancora non hanno avuto giustizia, mi unisco, anche a nome del mio Gruppo, all'appello della comunità ebraica affinché venga impedita qualsiasi iniziativa pubblica o privata a favore del detenuto Priebke, il quale non ebbe alcuna pietà verso i familiari delle vittime o delle persone che ha torturato in via Tasso e in tutti questi anni mai si è pentito e mai ha chiesto scusa. Roma è stata insignita della medaglia d'oro alla Resistenza e nessuno di noi può assistere in modo impassibile o distratto ai festeggiamenti di uno dei responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

dell'Aula del Senato, vi dovrebbero essere meno parole e più fatti. *(Commenti del Gruppo M5S).* Le proposte di legge sono già state presentate. Se non vi dovesse far garbo il cognome Scilipoti, sostituitelo, copiatele integralmente, ma chiedete al Presidente della Commissione finanze di calendarizzare queste due proposte

che sia stata calendarizzata. Questo significa che non ci sono né la voglia, né la disponibilità da parte di coloro che esercitano il ruolo di Presidente di Commissione di tenere in giusta considerazione il lavoro del singolo parlamentare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso *weekend* vi è stato un anniversario importante che è passato in sordina in queste Aule. Sono trascorsi dodici anni dal 21 luglio 2001, quando, in una Genova accesa dalle manifestazioni sorte intorno al G8 e attraversata della tragica notizia della morte di Carlo Giuliani, i reparti della Polizia di Stato fecero irruzione nella scuola Diaz, compiendo, secondo quanto riferito da Amnesty International, gravi violazioni dei diritti umani. Come si svolsero i fatti è cosa nota: dell'operazione si contarono 93 arresti e una quantità quasi analoga di feriti. Ribadisco che sono trascorsi dodici anni da quegli avvenimenti, ma le ragioni di fondo della nostra preoccupazione purtroppo non sono cessate, come dimostra il recente caso kazako della Shalabayeva: uno Stato e un potere politico che mostrano il lato più esposto di un insistito conformismo, affermando e smentendo, facendo melina e schermandosi dietro una ricostruzione fatta ad arte, fantasiosa e palesemente bugiarda, in cui neanche tre indizi fanno una prova. È noto che i processi sono stati ostacolati in ogni modo e non solo sono stati protetti i dirigenti imputati, tra cui ricordiamo i nomi di Gratteri, Caldarozzi e Luperi, rimasti in carica fino al luglio 2012 2012 e impediti nelle loro mansioni solo dal giorno successivo dell'interdizione confermata dalla Cassazione, ma anche la stessa funzionalità della polizia è stata messa a repentaglio, pur di garantire la massima forma di salvaguardia, assicurando addirittura promozioni ai maggiori imputati, a cominciare dai tre ora citati, anziché sospenderli come vorrebbero equanimità e buon senso, prima ancora di una esplicita normativa dell'Unione europea. Allora è bene ricordare in questa sede, signor Presidente, che di vuoto normativo si è trattato se nessun provvedimento è stato assunto. I giudici, infatti, hanno rimarcato l'assenza di una legge sulla tortura. Non risultano provvedimenti disciplinari per i 40 imputati riconosciuti responsabili per i falsi e gli abusi a Bolzaneto, quasi tutti coperti dalla prescrizione, né per i condannati che in teoria, passati i cinque anni, potrebbero tranquillamente ritornare come se nulla fosse mai accaduto. Molte cose, però, sono successe nel frattempo e non vogliamo rassegnarci alla retorica gattopardesca dei falsi riformismi, di chi vuol cambiare tutto perché nulla cambi: Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, i fatti di Chiomonte. Dopo le condanne di Bolzaneto niente è stato fatto, malgrado sia stato chiesto l'obbligo di indossare codici di riconoscimento sulle divise, cui i vertici e i sindacati di polizia sono inspiegabilmente contrari in uno Stato democratico; malgrado gli appelli per una legge sulla tortura, che preveda esplicitamente la non prescrivibilità; l'auspicata istituzione di un organismo indipendente per la protezione dei diritti umani, con compiti di ispezione, chiesta anche da Amnesty International, nonché la revisione della formazione del reclutamento delle forze dell'ordine.

Gli abusi trovano origine a monte, in un potere politico che viene meno ad una serie di precise responsabilità e che non ha esercitato la precipua funzione di controllo democratico sulla polizia, che ha così potuto tenere una condotta arrogante verso le vittime dei suoi abusi, e nei magistrati e nei ministri che si sono succeduti. L'ultima conclusione è la seguente. Nel libro di Giancarlo Livraghi «Il potere della stupidità», leggiamo che una forma diffusa di stupidità è l'incapacità di ammettere i propri errori e che il coraggio di dire «ho sbagliato» non è solo onesto, ma è anche un modo intelligente di ridurre il potere della stupidità. Sempre in questo libro Livraghi dice che la stupidità non sta nel commettere errori, ma nel non volersene accorgersene, nel non volerli capire, nel non saperli usare come una fonte di apprendimento. Cito allora una metafora di Popper, «Einstein e l'ameba»: mentre a causa dei suoi errori, Einstein sopravviverà proprio grazie ad essi. Qui si tratta di decidere se vogliamo essere Einstein o un'ameba.

Credo di non essere l'unico ad avere già rivolto più interrogazioni e, nel caso specifico, una al Ministro dei lavori pubblici per un'opera importante che riguarda il territorio della provincia di Varese, la tratta ferroviaria Arcisate-Stabio. Già un precedente sollecito da parte del Presidente dell'Assemblea non ha sortito alcun effetto. A tutt'oggi sono passati quasi sessanta giorni dalla richiesta e non abbiamo ancora avuto alcuna notizia riguardo ad interventi da parte del Ministro. facciamo presente che il territorio si sta attivando; al livello locale certamente c'è molta apprensione e preoccupazione, così come al livello regionale. Occorre mettersi in sincronia e considerare che in momenti come questi far vedere che l'istituzione è presente, anche semplicemente dando una risposta, è un messaggio importante che la politica deve dare ai cittadini. intervengo per rispondere alla sollecitazione del collega Scilipoti, che ci fa presente di avere presentato un disegno di legge sulla separazione tra banche d'affari e banche commerciali.

la mia collega Montevecchi, alla quale lei ha concesso un tempo assolutamente fuori dal Regolamento per esprimere il suo pensiero. Desidero dire che sono grato alle forze di polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, che rappresentano lavoratori

essere grato a chi, ripeto, lavoratore e in condizioni non facili, adempie al proprio compito per la tutela di tutti noi cittadini. come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta pomeridiana di giovedì 25 luglio 2013 si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri sui seguenti argomenti: